finestra"). Il Presidente della Repubblica, con lettera del 6 novembre 2023, ha informato che, con decreto in pari data, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha nominato giudici della Corte costituzionale il professor Giovanni Pitruzzella e la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi. Interpretando i sentimenti di quest'Aula, esprimo ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro.

apre una nuova finestra"). La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 14 novembre 2023, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni nella Circoscrizione estero e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide. Ve le ricordo: ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, senatore Francesco Giacobbe; ripartizione America meridionale, Mario Alejandro Borghese;

Signora Presidente, se dovessi dire chi è stato Mario Tronti direi che è stato un militante comunista. In questo, nella sua militanza, nel suo comunismo, c'è un'etica, c'è un'umanità che testimonia l'intera sua esistenza. La vicenda politica, intellettuale ed esistenziale di Tronti è tutt'uno con la sua appartenenza ad un popolo, ad una classe sociale che sta in basso, esclusa e diseredata, umiliata e offesa e che cerca riscatto ed emancipazione. «Io sento di essere, so di essere, uno dei terminali, infinitesimo, di una storia di lunga durata, storia millenaria, eterna, delle classi subalterne». Questo scrive nel testo che regala ad amici e compagni in occasione

me, giovane neolaureato, in una ricerca sull'operaismo politico. Non esagero se dico che Tronti era in qualche modo una figura leggendaria nel campo della sinistra; trent'anni prima, nel 1966, aveva pubblicato per Einaudi un libro destinato ad essere dirompente, «Operai e capitale», che divenne il manifesto dell'operaismo e che anticipò l'urgenza di tempi nuovi (il Sessantotto studentesco, il Sessantanove operaio), di cui quel testo divenne un riferimento. Tronti pone il tema di una rivoluzione nella ricerca sociale, nella prassi politica, nel linguaggio della politica; adotta uno stile letterario, quasi poemi in prosa, con frasi folgoranti, che sono continue scintille di pensiero. Il marxismo di Tronti mette apertamente in discussione lo storicismo, l'idealismo, il "progressismo" della tradizione comunista italiana. L'operaismo fu uno straordinario romanzo di formazione intellettuale, dirà Tronti, nato a contatto con la fabbrica e con il modello delle lotte operaie. Ci sono pagine molto belle in cui Rita Di Leo racconta l'incontro tra Raniero Panzieri e Tronti, che Panzieri definisce come "una specie di Marx italiano". Da quell'incontro nasce l'esperienza di «Quaderni rossi», da cui poi Tronti darà vita alla rivista «Classe operaia», operaia», con un nucleo di personalità unite da quello che sarà per sempre un legame indissolubile, "un'amicizia stellare" la definisce Mario rivolgendo lo sguardo ad Alberto Asor Rosa, Umberto Coldagelli, Massimo Cacciari, Aris Accornero, Rita Di Leo. *(Applausi).* Altri, tanti altri, si aggiungeranno tra gli affetti politici ed esistenziali di cui Mario andrà fiero.

Gli scritti di Tronti sono tradotti in molte università nel mondo. Sono innumerevoli e compongono una biblioteca ricchissima, una miriade di intuizioni, di suggestioni, un pensiero spesso vertiginoso che contiene un continuo insegnamento. "No, non si può accettare un ordine del mondo intriso di ingiustizie e le forme di vita che esso detta". Un pensiero con così tanta forza evocativa, e per questo capace di parlare a nuove generazioni di militanti, perché non ha paura di guardare in faccia l'altezza della voragine del tempo che viviamo. Tronti critica un presente senza storia e senza memoria, democrazie senza più partiti, senza più soggetti collettivi, dominate dalla demagogia, dove al posto del "popolo politico" c'è il "populismo antipolitico"; segnate dalla spoliticizzazione del potere politico e dalla neutralizzazione del conflitto sociale. Eppure la lotta di classe c'è ancora dice Tronti - e ci sarà sempre, fino a che ci saranno barriere sociali insormontabili. A noi, militanti di generazioni successive, Tronti ha insegnato questo: far vivere sempre, dando battaglia politica, il punto di vista della parte che storicamente si è chiamati a rappresentare; far vivere in forme nuove l'eredità storica del movimento operaio e popolare; aspirazioni, speranze, passioni di chi è sfruttato, nel mondo frammentato, precario, smarrito che viviamo. Tornare a fare società con la politica, perché la crisi della sinistra è tutt'uno con la crisi della politica. Tronti ci ha insegnato "l'autonomia del politico" e il valore del primato della politica, che non è autoreferenzialità, ma forza di un progetto sociale di cambiamento, perché quando la politica diventa subalterna allora è incapace di trasformare la società. Tronti sferza la sinistra a cercare nutrimento nella teologia politica, nel legame vivo, vitale, tra spiritualità e politica. «Rimane un mistero» scrive - «perché cristianesimo e comunismo non si siano incontrati. È una ferita della storia, un danno per l'umanità». Quell'umanità a cui Mario irriducibilmente appartiene. C'è scritto questo nella targa affissa sul muro della casa dove è nato: «Sono cresciuto nel quartiere Ostiense di Roma, una periferia urbana, i miei lavoravano ai mercati generali. Mio padre faceva lo scaricatore ed era comunista, mia madre aveva un banchetto. Gli operai e i tranvieri della sezione Ostiense del Pci [...] sono stati la mia scuola politica. Mi insegnavano che cos'era la lotta per la buona causa e le regole per ben condurla. Considero tutto questo il mio plusvalore umano». A Mario Tronti, politico, filosofo, comunista. *(Applausi)*.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi, a poco più di tre mesi dalla sua scomparsa, commemoriamo un senatore, un filosofo, un intellettuale fra i più originali che il nostro Paese abbia conosciuto; un uomo che è sempre stato di parte, ma che al tempo stesso si è sempre sentito di potere e dovere esercitare la critica anche nei confronti della propria parte; un uomo libero, uno spirito libero. La sua eredità è quella degli irregolari, dei pensatori che non possono essere incasellati in rigide appartenenze e categorie, ma che esplorano territori lontani, per molti aspetti opposti; e quando tornano dai loro viaggi, dai loro pellegrinaggi intellettuali, riportano una sintesi sempre nuova, provocatoria, mai banale. Tutto questo non vuole mascherare o edulcorare la realtà. Certo, Mario Tronti è stato un filosofo operaista, un filosofo comunista, un uomo profondamente e integralmente di sinistra. Gli oppressi, gli sfruttati, gli ultimi erano il suo punto di partenza, ma non erano il suo punto di arrivo, perché in mezzo c'era la politica, la politica che doveva rovesciare i potenti dai troni, la politica che doveva innalzare gli umili. Tronti credeva nella politica come mezzo per acquisire consapevolezza, emancipazione, potere da parte delle classi subalterne. Ma, proprio perché ha creduto nella politica, non ha mai prestato il fianco alle scorciatoie populiste, alle semplificazioni moralistiche o alle supplenze della magistratura e ha sempre espresso un'assoluta critica a ogni forma di populismo. Egli credeva - e, se ci permette, signor Presidente, noi con lui - nell'autonomia della politica, seguendo il pensiero di Max Weber e, dopo di lui, di Gramsci e di Carl Schmitt;

Tronti ha cercato, in particolare negli ultimi anni, chi fosse in grado di svolgere questa funzione, un compito che non poteva essere svolto dai cultori dell'organizzazione o, peggio, dalla ortodossia, ma da politici capaci di innovazione, dotati di capacità profetica, di cogliere il movimento reale della storia e di porsene alla guida. Di qui il suo profondo distacco da tutti i tentativi, anche i più recenti, di restaurazione di una sinistra identitaria, velleitaria, minoritaria; una sinistra totalmente priva di realismo politico. Signor Presidente, vorrei concludere proprio su questo concetto. Mario Tronti fu tra i primi, a proposito di capacità profetica, a capire che dopo il 1989, dopo la caduta del Muro, il mondo sarebbe stato più incerto, più instabile e più insicuro; insomma che non ci sarebbe stata la fine della storia, ma che, anzi, un Paese come l'Italia sarebbe stato chiamato ad assumersi responsabilità internazionali, come poi puntualmente è avvenuto. Nulla di più lontano dal pacifismo imbelle, dall'irenismo incosciente e inconcludente che attraversa, come una tentazione nascosta, pensieri e desideri di parte della sinistra nostrana. L'auspicio - e concludo - per noi che siamo rimasti su questi banchi, per noi senatori della Repubblica italiana, è custodire la memoria di Mario Tronti come un ammonimento: stare dalla parte degli ultimi, non solo con il sentimento ma con intelligenza, con competenza e con realismo politico.

Mario Tronti è stato un senatore apprezzato, rispettato e a cui giustamente oggi il Senato rende onore. Ma tutti sappiamo che la vita di Tronti e l'opera per la quale verrà ricordato non sono state certamente soltanto in quest'Aula. Mario Tronti è stato uno dei grandi intellettuali di un'epoca brillante e densa di grandi intelligenze, forse il principale e più ardito innovatore di un pensiero marxista che per lui non aveva nulla di ossificato, di dogmatico o di scolastico. Fu proprio la politica a costituire sempre il centro e l'asse della sua opera di filosofo e anche per una lunga fase della sua attività di militante negli anni straordinari delle riviste operaiste alle quali offriva un contributo impareggiabile: i «Quaderni rossi» di Panzieri, «Classe operaia» e poi, molto dopo, in una fase storica assai diversa, «Laboratorio politico». Tronti incarnava un modello di intellettuale molto distante da quello a cui siamo abituati oggi; un pensatore per cui l'intervento politico sulla realtà e la riflessione teorica erano inscindibili, non solo e non tanto perché l'obiettivo della sua ricerca era sempre e solo la modifica o il ribaltamento degli equilibri sociali, e soprattutto perché era a partire dalla ricerca sulla realtà della classe operaia del suo tempo che il suo pensiero traeva linfa. Nei giorni successivi alla sua scomparsa, Tronti è stato definito da più voci il padre dell'operaismo. Lo era davvero, ma il suo operaismo non consisteva nel pretendere di insegnare qualcosa alla classe operaia; al contrario, dagli operai e dalla loro composizione di classe, dalle loro esigenze, dalla loro conflittualità, Tronti voleva imparare e imparò. Capovolse la visione classica marxista mettendo al centro dello sviluppo non più le strategie del capitale, ma il conflitto operaio, che il capitale era poi sempre costretto a inseguire; non si inventò quel rovesciamento a tavolino, ma lo apprese di fronte ai cancelli delle fabbriche. Scoprì che la composizione di classe era cambiata, che era emersa la nuova figura che sarebbe poi stata protagonista del ciclo di lotte straordinario degli anni successivi (gli anni Sessanta e Settanta), osservando e partecipando ai conflitti reali. Non fosse altro che per questo, per questa capacità oggi scomparsa di imparare avidamente e con profonda passione politica dalla realtà, dovremmo tutti guardare a Tronti e alla sua generazione intellettuale come esempio a cui ispirarci; così come dovremmo imparare da un'altra eresia che vide Tronti tra i suoi pionieri: pur restando solidamente un uomo di sinistra e senza nulla concedere a quelle ambiguità teoriche oggi tanto in voga, Tronti fu tra i primi a studiare e a cimentarsi con pensatori lontani dalla sua posizione, senza farsene sedurre, ma neppure proibendosi per vincolo ideologico di metterne a frutto le intuizioni. Già in precedenza, ma poi negli anni più recenti, quando cominciava la crisi del movimento operaio e per la politica, in essa la sinistra, una lunga traversata nel deserto, le riflessioni di Tronti sull'elaborazione della sconfitta dimostrano tutta la grandezza della sua libertà di pensiero: quella capacità, cioè, di non escludere per fanatismo ideologico la possibilità di studiare e anche imparare da pensatori su posizioni opposte alle proprie, senza per questo smarrire la parzialità e il punto di vista di un pensiero radicale. una ricerca intellettuale, appunto radicale, che pure seppe accompagnare a un realismo politico, che muoveva dall'idea di spostare il conflitto nella politica e nello Stato. Anche questo mi pare un punto importante non solo nella produzione, ma anche nella biografia di Mario Tronti. Pochi possono essere definiti, più a buon diritto di lui, un padre del Sessantotto. Eppure, quando esplose una rivolta operaia che confermava molte delle sue intuizioni, quando un nuovo biennio rosso sembrava davvero colorare l'alba, ma forse era invece un annuncio del tramonto, Tronti rimase consapevole che, senza un forte e strutturato partito di massa, radicato nella società e attivo in Parlamento, a farne le spese sarebbe stata, prima di tutti, proprio la classe operaia. Il suo lavoro sull'autonomia del politico deriva proprio dalla percezione lucida della sconfitta che si era nel frattempo consumata e cerca nel politico una via per evitarne le conseguenze più dirompenti: per salvare il salvabile, potremmo dire. Il quadro sociale e politico di oggi, Presidente, è molto diverso da quello in cui maturarono gli elementi essenziali del pensiero di Tronti. Ma l'eredità dei veri grandi intellettuali consiste nel lasciare modelli e metodi che possono essere rimodulati in maniera feconda, anche a fronte di circostanze diverse. Questo ci lascia Mario Tronti: un modello di intellettuale e, soprattutto alla sinistra, un metodo che dovremmo essere capaci di riprendere. Per questo, e anche per questo, lo ricordo con grande affetto e, a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra, rivolgo ai suoi familiari, ai suoi compagni, ai suoi amici, il nostro saluto più caro.

quindi in due periodi storici completamente diversi: il primo, quello del Governo Amato, apre la strada al Governo tecnico del governatore Ciampi, in una legislatura durata solo due anni e che segna la fine della Prima Repubblica; il secondo periodo vede tre Governi di sinistra, dal 2013 e al 2018. Tronti è in ogni caso già presente nelle nostre enciclopedie, come la Treccani, per essere stato un fine intellettuale, attento alle questioni di sinistra, ma anche a quelle dell'area cattolica. Degno di nota il suo lavoro di intellettuale marxista, che legge e rivaluta Nietzsche e il suo pensiero nichilista e razionalista, cercando di comprenderlo nell'alveo filosofico della sinistra: cosa particolare, posto che si trattava di un filosofo che è sempre stato vicino al pensiero di destra. L'impegno di professore universitario, filosofo e intellettuale, lo ha visto porre il tema della classe operaia al centro delle sue attenzioni; tanto che, scrivendo testi come «Operai e capitale», ma anche fondando, assieme ad altri, la rivista «Classe operaia», ha alimentato e reso comprensibile ai più il pensiero, le rivendicazioni operaie e della remunerazione del lavoro rispetto al capitale. Erano gli anni in cui si pensava che la classe operaia potesse andare in paradiso. Ora in paradiso è andato lui, ma lascia sulla terra il suo pensiero, i suoi studi, la sua grande onestà intellettuale, un'eredità di cui possiamo beneficiare tutti. Va ricordato, infine, che il Senato ha acquisito la documentazione della sua vasta esperienza intellettuale attraverso la donazione di tutto il suo archivio nel 2022 e sarà questo, sicuramente, fonte per ulteriori studi. condiviso con il senatore Tronti la seconda delle due legislature in cui il collega ha fatto parte di questa Assemblea. sottolineare quanto coloro che sono intervenuti prima di me hanno illustrato della sua vita, del suo orientamento e della sua opera. La cosa che

volontà di proseguire nell'analisi che aveva sempre portato avanti nella sua lunga carriera di accademico, di intellettuale di filosofo, facendolo anche quando poteva essere scomodo. L'intervento che più mi restò in mente, che poi sono tornato a leggere una volta che ho saputo di questa commemorazione, è quello che lui chiese di fare il 24 ottobre 2017 - facile ricordare la data - nel centenario della Rivoluzione detta di ottobre, dove specificò che il 24 ottobre era la data del calendario giuliano perché in quello gregoriano era già

e anche poi quanto ne seguì, di cui denunciò altresì - usando anche la persona la parola crimini - i gravi problemi che da essa derivarono. Ovviamente io e il Gruppo che ho l'onore di presiedere non abbiamo condiviso le sue idee neanche in quella circostanza. Ma è stato interessante conoscere la

si erano seguiti, rinnovando quell'impegno politico che ha caratterizzato tutta la sua esistenza sia nell'Aula del Senato, per due legislature, sia al di fuori delle Aule parlamentari. il finale del suo intervento di quel 24 ottobre 2017 possa essere di insegnamento e possiamo condividerlo tutti. Nel terminare il suo intervento il senatore Tronti disse che egli continuava, anche in quel momento della sua carriera e della sua vita politica, a perseguire gli stessi fini di sempre sia pure in condizioni molto diverse da quelle che dall'inizio della sua carriera, anche solo nella precedente legislatura in cui era stato senatore, e probabilmente, anzi certamente - come diceva apertamente - in condizioni che lui non avrebbe voluto vivere. Disse che il fatto di continuare a portare avanti quegli stessi ideali sia pure con altri mezzi era un esercizio spericolato, ma entusiasmante.

in modo spericolato, ma entusiasmante, credo sia davvero un insegnamento per tutti noi. Anche per questo io sono lieto di salutare, a nome di tutto il mio Gruppo, i suoi familiari presenti e i suoi amici, nel ricordo comune di una figura che indubbiamente ha segnato la vita politica dell'Italia.

restando nell'attualità del dibattito, che per il senatore Tronti la parola pronunciata in Parlamento non era mai puramente tecnica, ma era un'arte parlamentare. Possiamo dire che per Tronti il parlamentare coincideva con «Parlare in Parlamento» di Vittorio Emanuele Orlando. La lezione di Mario Tronti potrebbe sintetizzarsi oggi come un testamento di fiducia per il Parlamento; un Parlamento non solo decidente, ma, prima ancora, un Parlamento pensante. ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, per aver fatto vibrare in quest'Aula la tensione ideale che ci ha trasmesso Mario Tronti nella lotta contro l'ingiustizia sociale, nel nome del lavoro, dei suoi dei suoi diritti e di un umanesimo militante.

la Commissione finanze e tesoro ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 132, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Il conferimento del mandato al relatore avverrà dopo l'acquisizione del prescritto parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti approvati nella seduta odierna. La Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di domani alle ore 9,15, quindi nella giornata di domani siamo convinti di poter concludere tutto l'*iter*.

intervengo sull'ordine dei lavori, per far notare ai colleghi e alla Presidenza, che inevitabilmente ha provveduto a far scorrere l'ordine del giorno, che siamo arrivati esattamente lì dove giovedì avevamo previsto che saremmo arrivati. E giovedì, con il presidente Patuanelli e con i Presidenti di tutti i Gruppi di opposizione, avevamo fatto queste previsioni non perché siamo diventati all'improvviso dei chiromanti, signora Presidente, perché era evidente che il lavoro che le Commissioni stavano

ascoltare con meno arroganza le ragioni dell'opposizione, in una fase delicata come questa *(Applausi)*, nella quale stiamo cercando semplicemente di rispondere ai mondi esterni. Dopo aver preso atto che la maggioranza non vuole emendare la legge di bilancio, nonostante le critiche durissime arrivate in questi giorni di audizioni e nonostante oggi si sia arreso all'evidenza anche il Ministro dell'economia, quello che stiamo cercando di fare è tenere insieme tutti i provvedimenti che hanno un impatto economico (vale per il disegno di legge cosiddetto proroga termini provando a evitare che fuori non si raccontino cose impossibili da attuare, per consentire a tutti i Gruppi parlamentari, compresi quelli a cui non sarà data la possibilità di emendare la legge di bilancio, di intervenire sugli altri provvedimenti. Come vedete, care colleghe cari colleghi, oggi siamo nella condizione di prendere atto che il tempo trascorso da giovedì alla giornata di oggi sul disegno di legge di proroga termini e sul disegno di legge sulla concorrenza è passato invano. Avremmo potuto lavorare e intervenire insieme su quei temi blindati

siete costretti a darci ragione. Noi restiamo qui, signora Presidente, aspettando che prima o poi la maggioranza prenda atto che lavorare con l'opposizione è utile per il Paese.

la scorsa settimana non si è tenuto nemmeno il rituale *question time*, perché - si diceva - sarebbe stata una settimana lunga, saremmo andati avanti fino a venerdì e avevamo tante cose da fare, tra cui la legge annuale la legge annuale sulla concorrenza e il decreto cosiddetto proroga termini. Avevamo in calendario un sacco di provvedimenti, per poi scoprire che alle ore 14 bisognava abbandonare l'Aula per andare a fare altro,

Oggi il Governo ci dice, in Commissione bilancio, che tutti i pareri sono contrari per assenza di relazione tecnica. È evidente, quindi, che la Commissione non ha lavorato in questi giorni per arrivare a darci dei pareri di merito sui profili economico-finanziari di quegli emendamenti, ma semplicemente ciò che ha fatto oggi poteva farlo giovedì scorso e giovedì e venerdì mattina avremmo potuto lavorare in modo ordinato sul disegno di legge annuale per la concorrenza.

per associarmi alle osservazioni che sono state formulate dai colleghi, che inevitabilmente ci inseriscono dentro un quadro di valutazione di carattere più generale, perché non possiamo non esprimere un grado di preoccupazione rispetto al ruolo e alla capacità con la quale il Parlamento viene chiamato in causa e può incidere. È evidente che le modalità con le quali il Governo, in diverse circostanze (ne vorrei citare solo due a titolo esemplificativo), tende ad esautorare l'azione fondamentale del Parlamento, vengono complicate da questo tipo di programmazione e da questo tipo di attività che è stata messa in campo, con il risultato di dare l'impressione, l'immagine o la rappresentazione di un'Aula svuotata quando questo non è, o quantomeno non lo è dal punto di vista dei rappresentanti dell'opposizione, che avevano già formulato questo tipo di preoccupazioni la scorsa settimana e che ora si trovano inevitabilmente chiamati a dover confermare lo stato della loro previsione. Rispetto alla tendenza ad immaginare che il Parlamento sia un luogo di ratifica, ci sono due elementi che mi permetto di portare alla sua attenzione e all'attenzione dei colleghi: il primo - ne abbiamo già discusso in altre circostanze il rischio di svuotare il Parlamento rispetto a una questione significativa ed importante qual è quella dell'annunciato accordo internazionale fra Italia e Albania in materia di immigrazione; il secondo, che abbiamo appreso oggi sulla stampa,

in molte discussioni in questi ultimi anni, cioè la cosiddetta applicazione o revoca del protocollo sulla cosiddetta Via della Seta. Immaginare che una questione di questa natura possa essere archiviata e derubricata al rango di una questione amministrativa una volta di più, interpretare in maniera erronea il ruolo di questo Parlamento. *(Applausi)*. Allora, se alla pervicacia del Governo aggiungiamo anche la confusione da parte della maggioranza, c'è motivo per esprimere preoccupazione.

il disegno di legge n. 795, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, è stato modificato in Commissione attraverso l'approvazione di numerosi emendamenti che hanno inteso ampliare il perimetro del provvedimento. La legge annuale per il mercato e la concorrenza, definita dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ha come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private e la tutela dei consumatori. In aggiunta a ciò, l'adozione di leggi annuali sul mercato e la concorrenza è un contenuto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con precise scadenze; in particolare, per il 2022 il PNNR ha individuato come necessarie le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2. Il contenuto del disegno di legge annuale è di per sé eterogeneo, dato il carattere finalistico del provvedimento, che costituisce proprio l'elemento comune a tutte le disposizioni. Venendo all'articolato, l'articolo 1 del disegno di legge, modificato in Commissione, modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni due anni anziché annualmente, precisando che essi devono essere predisposti dall'impresa di maggiori dimensioni con riferimento al trasporto di gas naturale, tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete. Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale presentati ogni due anni da Terna, si fissano i seguenti termini procedimentali: sessanta giorni per l'espressione dei pareri da parte delle Regioni e delle Province autonome interessati; sei mesi dalla presentazione del piano per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'ARERA; diciotto mesi, comprensivi della valutazione ambientale strategica, per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali termini decorrono nuovamente, ridotti della metà, qualora Terna presenti integrazioni al piano già trasmesso. L'articolo 2, non modificato dalla Commissione, reca alcune disposizioni volte ad attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, anche mediante la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione nell'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico SpA. L'articolo 3, non modificato dalla Commissione, inerisce al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (*cold ironing*) e al proposito offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA. L'articolo 4, introdotto dalla Commissione attraverso l'approvazione di un emendamento dei relatori, è volto a garantire che i decreti ministeriali coi quali vengono definite le modalità di applicazione in ambito ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, siano adottati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Tale precisazione è funzionale ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento interno ai principi europei in tema di sicurezza del trasporto ferroviario, considerato che in ambito ferroviario qualsiasi norma nazionale che risulti non conforme e/o ridondante rispetto alle norme europee vigenti, quali le specifiche tecniche di interoperabilità e i metodi comuni di sicurezza (CSM), deve essere abrogata, pena l'avvio di una procedura di infrazione. Per analoghe esigenze di garanzia e certezza del diritto si prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo, in forza del quale i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono predisporre, sulla base di un'analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati lungo la rete ferroviaria. Tali adempimenti devono essere sempre effettuati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e interoperabilità del trasporto ferroviario. Per questi motivi, ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento dei titoli formativi posseduti e delle mansioni ricoperte. L'articolo 5, introdotto dalla Commissione, consente agli aspiranti conducenti dei mezzi di trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in Province diverse da quelle di residenza nel caso in cui in queste ultime non siano previste sessioni d'esame. L'articolo 6, inserito dalla Commissione, disciplina le modalità di pubblicità delle informazioni relative ai contributi che i produttori di apparecchiature elettroniche ed L'articolo 7, introdotto durante l'esame in sede referente, apporta modifiche al codice della nautica da diporto novellando la disciplina della mediazione con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e ai più rigorosi livelli di formazione professionale. Le principali novità introdotte dal nuovo testo sono la specificazione che il mediatore professionale, per godere e sottostare al relativo statuto giuridico, deve svolgere l'attività descritta nel comma 2 e con le caratteristiche ivi indicate, anche in chiave occasionale o temporanea, fermo restando il requisito dell'indipendenza da entrambe le parti dell'affare; le esplicitazioni del rinvio alla normativa euro-unitaria sul mutuo riconoscimento dei titoli abilitativi e alla normativa di attuazione del Testo unico sull'immigrazione, sul riconoscimento dei titoli abilitativi per i cittadini dei Paesi terzi; l'individuazione del Ministero delle infrastrutture come come Autorità nazionale competente per la figura professionale del mediatore della nautica da diporto. L'articolo 8 prevede l'adozione di un decreto del

In virtù di un emendamento approvato dalla Commissione, si stabilisce che nei contratti stipulati a distanza il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le disposizioni contrattuali trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile. L'articolo 9, inserito durante l'esame in sede referente, reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

L'articolo 10, introdotto in sede referente al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità senza pregiudizio per la salute pubblica prevede e disciplina l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, dei parametri attualmente vigenti, limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 1). Scaduto il citato termine, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti Sono inoltre apportate modifiche alla legge n. 36 del 2001, in particolare al fine di prevedere il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nelle funzioni in materia di L'articolo 11 interviene sulla modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein 2006/123/CE, e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo le linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano le procedure selettive (comma 3). L'articolo 5 dispone inoltre che continuino ad avere efficacia fino al termine previsto del relativo titolo le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall'articolo 181, commi 4-*bis* e del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre del 2020 e che, allo stato, non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate, salvo rinuncia dell'avente titolo, in virtù di una modifica apportata dalla Commissione e salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela Inoltre, nelle more della preparazione dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6). Con il comma 8, inserito in sede referente, si proroga proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'operatività della norma introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma in oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie e stagionali,

dell'Istituto comprensivo «Sacro Cuore» di Napoli, che assistono ai nostri lavori.

e la concorrenza è stato fatto un lavoro importante da parte della Commissione: il testo è entrato con dieci articoli e ne esce con ventuno. Abbiamo fatto un lavoro molto ringrazio il sottosegretario Bitonci per la collaborazione, così come ringrazio il presidente De Carlo, tutti i commissari e gli Uffici. Riprendo da dove ha lasciato il mio collega, ossia dall'articolo 12, che è stato modificato in sede referente che include, nelle motivazioni che legittimano le vendite di liquidazione, anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte e di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile. Il comma successivo, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell'impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in Comuni diversi. In particolare, la norma consente all'impresa di presentare in via telematica allo sportello unico attività produttive dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e le indicazioni di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP riceve a sua volta e trasmette la comunicazione con modalità telematica a tutti i SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi. La relativa documentazione è tenuta a disposizione dell'autorità di controllo per due anni oppure sul relativo sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione. L'articolo 12, al comma successivo, cioè al comma 3, reca, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. In particolare, nel confermare quale principio generale dell'ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza limiti contingenti o altri vincoli, estende le casistiche in presenza delle quali è consentito fare eccezione a tale principio, con riferimento alla salvaguardia della sicurezza o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tale finalità, le Regioni, le Città metropolitane, e i Comuni possono, senza discriminazione tra gli operatori, disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico, culturale o commerciale, laddove viene prescritto che le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza vincoli inerenti al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, facendo salva la facoltà concessa, ai sensi della lettera *b)*, agli enti territoriali di imporre limitazioni all'insediamento di determinate attività. Il medesimo articolo 12, che è molto complesso, inserito in sede referente, integra i princìpi e i criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le Regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la libera realizzazione del settore del commercio e della pertinente normativa sui beni culturali e del paesaggio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori, senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico, culturale o commerciale, anche tramite la costituzione di specifici albi. L'articolo 13, inserito dalla Commissione, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione l'applicazione agli utenti di condizioni diverse in ragione del fornitore di provenienza. interverrà anche il Governo con un emendamento che è stato presentato in Aula. L'articolo 14, introdotto in sede referente, prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo per il professionista di inviare un avviso al consumatore giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta. L'articolo 15, introdotto durante l'esame, interviene modificando la disciplina normativa riguardante la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. In particolare, introduce, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea in materia di igiene dei prodotti alimentari, la previsione che le fasi del lavaggio e dell'asciugatura non si applicano ai prodotti di quarta gamma, il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge già all'interno di siti chiusi, ossia secondo specifiche procedure automatizzate in ambienti a clima controllato e dotati di livelli di filtrazione dell'aria adeguati ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate. È inoltre stabilito che il Masaf, di concerto col Ministero della salute e il Mimit, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, individua le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di quarta gamma compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.

all'Autorità garante delle comunicazioni delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione. L'articolo 18 non è stato modificato. L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni ammesse ai sensi dell'articolo 4, comma 7, sono sia dirette che indirette e riguardano, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura del mercato, anche le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori. L'efficacia di tale previsione viene condizionata alla pubblicazione sulla «*Gazzetta Ufficiale*» di linee guida, con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico, che dovranno essere adottate dal Mimit entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle disposizione in esame. L'articolo 20, anch'esso inserito in sede referente, modifica l'articolo 180, prevedendo che l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore, svolta dalle società di gestione collettiva, esercitata anche per effettuare la concessione di licenza e autorizzazione per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva. I criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, per ciascuna categoria di diritti intermediati, saranno individuati con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. modifica la legge sulla concorrenza 2021, differendo il termine per l'adozione di disposizioni modificative ed integrative del regolamento, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad un'autorizzazione paesaggistica semplificata nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, la fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati, introdotti mediante norme di legge. *(Applausi)*.

Signor Presidente, onorevoli senatori, tutelare le imprese italiane, le partite IVA, garantire i diritti dei cittadini consumatori, liberare e mettere in circolo le energie migliori del mondo produttivo italiano; sono questi gli obiettivi ambiziosi a cui mira il disegno di legge per il mercato e la concorrenza, che è oggi all'esame dell'Aula. La concorrenza è il cuore pulsante di qualsiasi economia sana perché stimola l'innovazione, riduce i costi per i consumatori, migliora la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. La concorrenza favorisce la crescita economica perché promuove l'ingresso di nuovi attori nel mercato ed incoraggia le imprese a diventare sempre più competitive. Il provvedimento di legge che ci apprestiamo a votare si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un duplice motivo. In primo luogo perché l'approvazione annuale di una legge sulla concorrenza rientra negli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. In secondo luogo perché il disegno di legge contiene una serie di norme necessarie per il raggiungimento di alcuni obiettivi previsti dal PNRR. Tra questi provvedimenti ci sono sicuramente quelli che riguardano il potenziamento e lo sviluppo della rete elettrica nazionale e la norma per la promozione dell'uso dei cosiddetti contatori intelligenti, con l'obiettivo di favorire il risparmio energetico e di contenere il prezzo dell'energia elettrica. Il disegno di legge affronta e risolve l'annosa questione dei commercianti ambulanti che rischiavano di finire stritolati dalla direttiva Bolkestein. Finalmente, grazie al grande lavoro portato avanti dalla Lega e in particolar modo dal sottosegretario Massimo Bitonci, è stata trovata una soluzione positiva in sinergia con le associazioni di categoria, che dà certezze e che tutela concretamente migliaia di piccoli imprenditori che svolgono attività fondamentali nei mercati dei nostri Paesi. Il rinnovo in via eccezionale per dodici anni delle attuali concessioni e i criteri premiali fissati per i bandi delle future concessioni, che avranno una durata di dieci anni, sono la chiara dimostrazione di come la Lega ha saputo difendere con successo 180.000 aziende italiane, senza cedere alle assurde imposizioni di Bruxelles. *(Applausi)*. che il Governo di centrodestra userà la stessa determinazione per difendere le spiagge italiane e gli imprenditori balneari dalle follie della direttiva Bolkestein. legge concorrenza introduce anche una serie di norme volte a rafforzare il ruolo e il potere dell'Antitrust, per garantire che le leggi siano applicate correttamente e per garantire che le pratiche sleali e gli abusi di posizione dominante siano sanzionati in maniera efficace. Il disegno di legge sulla concorrenza è stato arricchito e migliorato grazie al lavoro che abbiamo fatto in Commissione e grazie alla positiva interlocuzione che abbiamo creato con il Governo, in particolar modo con il sottosegretario Bitonci, al quale vanno i nostri ringraziamenti. proposito vorrei porre l'attenzione su alcuni dei tanti emendamenti presentati dalla Lega e da tutta la maggioranza, che hanno contribuito a migliorare sensibilmente il testo di legge e a trovare soluzioni concrete alle giuste esigenze segnalate dalle associazioni di categoria. Penso agli emendamenti migliorativi sulla questione degli ambulanti, penso all'emendamento sulla tutela delle botteghe storiche, che finalmente dà agli enti locali una serie di strumenti per salvaguardare queste attività, che rappresentano un patrimonio culturale, economico e sociale di fondamentale importanza per le nostre comunità. Penso all'emendamento che regola e tutela i prodotti ortofrutticoli coltivati nelle *vertical farm*. Penso all'emendamento che garantisce maggiore trasparenza sulla tutela del diritto d'autore oppure all'emendamento che semplifica l'accesso alla professione di autotrasportatore. Penso infine all'emendamento che recepisce l'indicazione dell'Antitrust che mette fine alla discriminazione tra gli utenti di telefonia mobile che ricevono offerte discriminatorie sulla base dell'operatore di provenienza. Il disegno di legge concorrenza, grazie a questi importanti correttivi,

di provenienza. Il disegno di legge concorrenza, grazie a questi importanti correttivi, si inserisce pienamente nel solco di altri provvedimenti fin qui adottati dalla maggioranza e dal Governo di centrodestra, che dimostrano in maniera chiarissima la nostra attenzione e la nostra volontà di aiutare, supportare e promuovere lo sviluppo delle imprese e del mondo produttivo italiano. È in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare, tagliando la burocrazia, semplificando e rimuovendo gli ostacoli che frenano la crescita economica, per costruire un'Italia più forte, più competitiva e più giusta.

la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha un fine molto chiaro, semplice, ma estremamente determinante: rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, aprendo allo sviluppo della concorrenza e garantendo la tutela dei consumatori. Si tratta di una legge annuale, perché il mercato non è un'entità astratta e immobile, alla quale basta una registrata di tanto in tanto per essere regolato. Il mercato è vivo, attivo, frenetico, soggetto ai cambiamenti di una società aperta e contaminata dallo sviluppo

e ottenere prodotti di migliore qualità a prezzo più basso. Per fare ciò non si può che partire dal regolamentare e innovare un mercato, quello energetico, che i tempi moderni richiedono essere sempre più un mercato volto alla tutela ambientale, al rinnovabile, al virtuoso. Ci aspettavamo in questo disegno di legge che la tematica energetica fosse affrontata con l'attenzione che merita e con quel coraggio di innovare che anche gli ultimissimi disastri naturali rimarcano come necessario e non più rinviabile. Invece, le misure energetiche presentate nel disegno di legge hanno un impatto quasi nullo su questo settore strategico per la concorrenza, per la produzione e per i consumatori, cioè aziende e famiglie italiane. Mancano strumenti che, a nostro avviso, sarebbero indispensabili per consentire a imprese e consumatori di adottare comportamenti virtuosi. I soli contatori intelligenti di seconda generazione non bastano: sono un primo passo, ma da soli non sono sufficienti. Serve un coinvolgimento diretto di imprese e consumatori, il cui ruolo nello sviluppo e nel risparmio energetico è critico e dev'essere valorizzato e potenziato con strumenti legislativi efficaci e inclusivi. e inclusivi. È quanto mai evidente poi che in questo disegno di legge non si è fatto praticamente nulla per garantire alle imprese maggior concorrenza nell'offerta di energia elettrica e gas naturale. La mancata proroga dell'entrata in vigore del regime di libero mercato per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici determinerà costi insostenibili per le famiglie italiane, che già devono fare i conti con l'inflazione e una situazione internazionale che, in termini di fornitura energetica, lascia poco spazio alla speranza di risparmio. I costi per le famiglie italiane aumenteranno già a partire dal prossimo anno. Da questo disegno di legge traspare l'assenza di una visione strategica sulla politica energetica di medio e lungo termine, una strategia che porti il Governo a investire nella diversificazione delle fonti energetiche, nel potenziamento delle infrastrutture e nella costruzione di una nuova capacità di rigassificazione e nel rafforzamento di quella esistente. Approvare oggi questo disegno di legge che non innova nulla e non arreca modifiche amministrative efficaci vuol dire aver perso l'ennesima occasione per offrire al Paese, alle aziende e ai cittadini cambiamenti sostanziali, che avrebbero potuto avere un impatto determinante nella vita quotidiana. *(Applausi)*. Dovremo aspettare un altro anno per sperare di poter innovare settori su cui dovevamo mettere le mani oggi, ma ad essere onesti il futuro non lascia intravedere nulla di buono; anzi, sembra che si vada verso un peggioramento costante. concorrenza e innovazione, innovazione vuol dire investire anche sui nostri cervelli in fuga e sui lavoratori specializzati che ogni anno abbandonano il nostro Paese, proprio perché il nostro mercato del lavoro non è concorrenziale. E qual è la risposta a queste carenze? Il Governo intende tagliare i benefici fiscali per quanti decidono di ritornare in Italia: un altro schiaffo al contributo dell'innovazione che i nostri connazionali di rientro potrebbero offrire al nostro Paese. Su questo, signora Presidente, e sulla difesa di una norma che - come indicato la scorsa settimana nel rapporto Migrantes - ha fatto tornare in Italia il doppio dei lavoratori rispetto ai decenni precedenti, annuncio fin d'ora che daremo battaglia in Commissione. Tornando al disegno di legge sulla concorrenza, le altre misure che sono riportate nel provvedimento oggi in al nostro esame, più che una rimozione degli ostacoli per le aperture del mercato assomigliano a una chiusura, alla conservazione di uno *status quo* che non fa bene né alle imprese, né ai consumatori. I settori su cui si è intervenuti poco e male sono una parte infinitesimale di quelli attesi. Le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non sono state recepite (anzi, sono state ignorate), così come sono state ignorate quelle della Commissione europea su temi importanti come le concessioni balneari, che sono scomparse dal disegno di legge. Ancora una volta, non si mette mano a una questione delicata, nonostante il richiamo del Capo dello Stato all'indomani dell'approvazione del decreto milleproroghe e i richiami della Commissione europea. Si è scelto di non scegliere e nel caso dei *dehors*, addirittura, di prorogare per un anno provvedimenti emergenziali studiati per il rilancio economico del post-pandemia. Fino a dicembre del 2024 saranno in vigore il regime semplificatorio e la possibilità di utilizzare temporaneamente il suolo pubblico senza pagare il canone di occupazione: è un provvedimento che aveva senso nell'immediato post-pandemia, ma non ora. Noi siamo favorevoli a concedere maggiori opportunità di impresa e sviluppo in tutti i settori, inclusi quello così nevralgico dell'ospitalità, ma questo va fatto questo va fatto sempre nel rispetto di tutte le parti e soprattutto nei confronti di chi vuole cominciare una nuova attività e vuole accedere al mercato e potersi trovare nelle stesse condizioni dei competitori, nel rispetto delle regole della concorrenza.

nonostante la vicenda abbia chiari risvolti dal punto di vista della concorrenza e della libera impresa. Le licenze nuove, infatti, sono limitate e quelle temporanee sono bloccate solo a chi già le detiene. Che definizione di concorrenza dobbiamo trovare per giustificare queste scelte? scelte? Il provvedimento in esame non apre ad opportunità, ma spesso le blocca lasciando spazio solo a chi è già in attività o detiene concessioni o licenze. Anche in quel caso, dove alcune chiusure potrebbero essere condivisibili, si è intervenuti sopra le righe in modi che non faranno altro che aprire a nuove opportunità di scontro con l'Europa. Onorevoli colleghi, signor Presidente, la realtà è che il disegno di legge in esame è peggiorativo di uno *status quo* che richiedeva interventi forti, diretti e soprattutto efficienti, per garantire quello che questa legge contiene nel suo stesso nome: la concorrenza. Nulla di ciò che è contenuto in questo testo dà un impulso al nostro mercato. Io e i colleghi senatori del Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti al testo in esame in Aula. Signor Presidente, tramite lei mi rivolgo ai colleghi di maggioranza perché riflettano e, prima di votare, possano pensare all'interesse del Paese per cogliere l'opportunità di apportare miglioramenti al testo in esame. In conclusione, signor Presidente, mi permetta di affermare che, se non creiamo le basi per quella concorrenza sana che porta innovazione e stimola l'impresa e la produzione, non aumenteremo posti di lavoro, non creeremo condizioni economiche favorevoli per imprenditori e famiglie, non daremo impulso neanche alla ricerca di nuovi mercati nel mondo per continuare a puntare su uno dei settori di maggior successo dell'economia italiana, l'*export*. In poche parole, perderemo un'altra occasione importante, purtroppo una delle tante, per poter contribuire al benessere economico di questo nostro bellissimo Paese.

abbiamo ascoltato l'ennesima previsione di grigiore e di mancato sviluppo che sentiamo da più di un anno a questa parte. Peccato che da più di un anno a questa parte tutti gli indicatori economici e di sviluppo dicano cose diverse,

in cui si legge infatti che la legge per il mercato e la concorrenza deve avere cadenza annuale, perché è essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della nostra legislazione al fine di verificare che permangano tutti i vincoli normativi al gioco competitivo e al funzionamento efficiente dei mercati. Il piano prevede una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza dal 2021 al 2024; il disegno di legge per il 2022 dev'essere approvato entro il 31 dicembre 2023

Ministero delle imprese e del *made in Italy* stanno tutti procedendo in modo deciso, ma anche perché stiamo rimuovendo tutti quegli ostacoli regolatori che impediscono l'apertura dei mercati, per promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori. Questi sono che possono dare al nostro Paese un'immagine nuova, diversa, di Stato aperto alla libera competizione tra le imprese, con un approccio quindi volto alla creazione di occupazione e di crescita, esattamente il contrario di quello che

per eliminare gli ostacoli alla concorrenza nei servizi pubblici locali, nel trasporto pubblico locale, nella distribuzione del gas e dell'energia idroelettrica, nella ricarica elettrica e nei rifiuti - è l'Unione europea che ce lo dice, quindi anche su questo mi sembra che ci siamo messi molto bene la mano sulla coscienza ma anche degli impegni assunti per la liberalizzazione dei mercati al dettaglio dell'elettricità e del gas e per ridurre il numero dei giorni necessari per avviare un'impresa. Stiamo cambiando l'Italia, la stiamo semplificando e la stiamo aprendo. L'obiettivo è quello che questo Governo sta dimostrando di saper perseguire, cioè semplificare e velocizzare le procedure burocratiche e migliorare le normative di settore. È quello che ci hanno chiesto le imprese, i consumatori e i cittadini, per essere più competitivi in un mondo sempre più globalizzato e pieno di tensioni ed è quello che avevamo promesso ai nostri elettori.

perché accanto alla concorrenza, che presuppone ovviamente, come abbiamo detto fino adesso, l'eliminazione di tutte le posizioni, anche odiose, dominanti, abbattendo i monopoli, affinché vengano migliorati ed efficientati i servizi,

uno Stato che voglia considerarsi autenticamente sovrano deve necessariamente detenere la proprietà delle reti delle infrastrutture nei settori di rilevanza strategica, tutelando l'interesse nazionale. Non c'è contraddizione tra concorrenza e interesse nazionale, non c'è contraddizione tra libertà di impresa e rilievo di *asset* strategici. *(Applausi)*. Questo lo dico perché spesso, nella recente storia del nostro Paese, tutto questo non è accaduto e lo ricorderemo perché è importante che,

popolazione, con tutto quello che è stato scritto e fatto in questi anni. La stessa Europa ci ricorda fondamentalmente che, al di là della libera concorrenza, necessario che all'apertura di fette di mercato ci sia la consapevolezza di rendere impossibile e di minare la sovranità degli Stati membri e degli assetti strategici e degli interessi nazionali di quegli Stati. Questo è quello che stiamo facendo. Ricordate, cari colleghi, quando in Italia si veniva a fare *shopping*? Si venivano a comprare *asset* strategici di interesse nazionale, in quanto il nostro era l'unico Paese che non tutelava ciò che era fondamentale per avere la propria identità, la propria autonomia, la propria indipendenza.

le quali andavano dall'elevato livello dei costi sostenuti e dal loro incerto monitoraggio alla scarsa trasparenza connaturata ad alcune delle procedure utilizzate. Tutto questo fa rima con Romano Prodi, non so se questo ricorda qualcosa a qualcuno, a proposito di mettersi una mano sulla coscienza. Noi non siamo così, così, non ci siamo formati in questo modo, anzi pensiamo ancora che, pur accettando la libera concorrenza, bisogni proteggere gli interessi nazionali, che non sono astratti, ma sono quelli dei cittadini, delle categorie e degli imprenditori. Abbiamo fatto ancora un esempio, ma anche su questi esempi, la differenza è che noi siamo orgogliosi dell'emendamento che abbiamo presentato anche grazie ai nostri senatori di Fratelli d'Italia,

tasse, perché in città turistiche e artistiche come Roma o come tante città d'Italia, come tanti Comuni e tanti borghi, sia possibile anche bersi un caffè, mangiare una pizza, fare colazione stando a contatto con la storia, con la cultura e anche con la strada, perché no? Per noi non è una vergogna, è un vanto quello che abbiamo fatto e lo rivendichiamo con grande orgoglio, perché siamo diversi, non ci inchiniamo di fronte ai poteri forti, non facciamo privatizzazioni che fanno gli interessi di qualcuno tranne quelli del popolo italiano. Facciamo sintesi tra le varie necessità, nell'interesse dei nostri cittadini. Questa è la nostra concorrenza, questo è l'impegno per la sovranità nazionale.

per alcuni territori, a discapito di altri. Vorrei concentrarmi su alcuni aspetti, valutata l'entità anche della discussione generale, in cui altri aspetti saranno discussi da altri miei colleghi e oggetto anche di dichiarazione di voto. A proposito del tema delle antenne e dei campi elettromagnetici, è chiaro che noi tutti abbiamo un'esigenza, quella di dare un'idonea copertura al Paese, da Sud a Nord, dalle aree più popolate a quelle interne, perché fare impresa in un'area interna o in campagna presuppone di potersi collegare con il mondo con le stesse modalità garantite alle aree maggiormente servite.

Siamo passati dal canone unico a procedure semplificate che fanno sì, in assenza di un piano comunale di installazione, che possano essere messe in qualsiasi luogo si valuti più opportuno da parte della compagnia, purché abbia la disponibilità del terreno del soggetto concedente. Ciò significa che alcune persone si trovano, dalla mattina alla sera, antenne sopra la testa, con effetti importanti non tanto di salute pubblica, ma anche rispetto al fatto che, quando questo avviene in aree fortemente popolate, si generano anche fenomeni che riguardano la proprietà immobiliare

Chiediamo però che questa pianificazione avvenga su base comunale e territoriale, perché si possano valutare le esigenze. I territori non sono fatti solo di aree densamente popolate, ma di località, di frazioni e di campo aperto e molto spesso capita che nelle nostre aree interne abbiamo il segnale solo nei capoluoghi, dove c'è una concentrazione di antenne, ma poi non le troviamo nelle

almeno anche una località con meno densità e con meno istanze possa essere servita, perché anche quelle persone hanno il diritto di potersi connettere con il mondo.

la pianificazione che faccia sì che non ci siano luoghi e persone di serie A e luoghi e persone di serie B, tra centri urbani e aree interne *(Applausi)*, con la salvaguardia delle persone. La stessa cosa la diciamo sui *dehors* e sui suoli pubblici. Abbiamo una norma nata in una condizione emergenziale che si proroga di anno in anno. E noi domandiamo: ma quale imprenditore può tarare la sua attività e la sua impresa di anno in anno, valutando condizioni contingenti e legate alla proroga di un provvedimento di fine anno? Nessuno lo può fare. Allo stesso tempo, anche noi siamo favorevoli al fatto che si possa operare con le imprese e si possa avere anche il giusto ampliamento dei suoli pubblici dati in concessione, ma anche nel rispetto di una concorrenza tra le imprese. Non tutti, infatti, possono avere un suolo pubblico a disposizione, non tutti possono avere spazi alla pari di altri, per cui ci sono luoghi che, per loro connotazione, si prestano ad avere grandi spazi di suoli pubblici e altri che non lo consentono. L'effetto è che, se ci si espande a dismisura nei primi luoghi, si penalizza chi svolge attività in altre parti,

perché molto spesso, soprattutto nelle aree interne e anche in quelle turistiche, accade che vi sia un eccesso di suoli pubblici nel periodo turistico, ma difficoltà a prendere un caffè quando il periodo turistico cessa. Un piano di gestione dei suoli pubblici a livello comunale dovrebbe e potrebbe consentire che ci sia sempre un'attività aperta, qualsiasi giorno dell'anno. Per questo, non siamo contrari

degli ambulanti, che molto spesso nelle aree interne sono l'unico presidio di commercio per l'acquisto di talune tipologie di prodotti. C'è infatti stata una desertificazione del commercio nelle aree interne, quotidianamente, con una sequela di attività che chiudono, facendo sì che i residenti abbiano difficoltà nell'approvvigionarsi di quelle merci e di quei materiali, se non ricorrendo al sistema

tutto sia dovuto, anche in queste aree. Per poter vivere in un'area interna, però, devono essere garantiti i servizi. E qui arriviamo alla norma che prevede una ricognizione annuale da parte dei Comuni, con tutta una serie di elementi e penalizzazioni,

È questo che noi chiediamo, perché i nostri Comuni non ce la fanno più. Io parlo da amministratore locale. I nostri Comuni non ce la fanno più a correre dietro ad incombenze su incombenze, che poi si sommano a tagli su tagli. Penso al taglio sul sistema sanitario e sociale, che oggi appesantisce i nostri bilanci e fa sì che i nostri comuni si siano surrogati a fare quello che deve fare lo Stato. *(Applausi**).* Lo facciamo con piacere e con onore, ma abbiamo il bisogno e l'esigenza di avere la nostra autonomia anche dal punto di vista decisionale, che non può prescindere dalla capacità economica che i nostri bilanci devono avere e che, con questi provvedimenti, anche questa volta viene tagliata.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge che stiamo affrontando nella seduta di oggi tocca temi cruciali, intesi a favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. La tutela e la promozione della concorrenza sono elementi essenziali per sostenere le imprese, per proteggere gli interessi dei consumatori e per ampliare l'opportunità dei cittadini di accedere equamente al mercato. È quindi sconcertante assistere come, anche in questo provvedimento legislativo, non sia stata presa in considerazione la sostenibilità ambientale. In un contesto economico e di mercato stravolto dalle guerre, dai prezzi, dalla crisi climatica e dalle tensioni sociali, dove si richiedono nuovi modelli di sviluppo per accrescere la competitività nazionale, il Governo italiano continua imperterrito a proporre soluzioni obsolete alle nuove sfide che si presentano e proprio non vuole cogliere le opportunità economiche già tracciate dalle politiche energetiche ambientali a livello sia internazionale sia europeo. Eppure l'urgenza di adottare nuove misure che tutelino l'eccezionale patrimonio economico dell'Italia è sotto gli occhi di tutti. Urgono misure economiche e strutturali che, da un lato, promuovano l'innovazione e con essa la competitività delle imprese e, dall'altro, rappresentino un potente antidoto alla crisi climatica. I mezzi esistono, ma il Governo non li mette a terra. L'Italia sta subendo enormi danni economici a causa della crisi climatica. Gli ultimi dati Eurostat parlano di 36,5 miliardi dal 2010 al 2020, con una media di oltre tre miliardi e Il nostro Paese è ormai regolarmente colpito da eventi climatici estremi; penso solo alle immagini devastanti degli ultimi giorni in Toscana, ma anche in Lombardia e nella mia Regione, il Veneto. Penso però anche a tutte le altre Regioni precedentemente colpite. Ancora oggi, nel 2023, dobbiamo vivere nell'incubo di perdere persone care. Per sopperire a questa enorme mancanza da parte del Governo italiano rispetto a un'economia sostenibile, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra stiamo cercando di accelerare la discussione di una legge quadro sul clima, che possa assicurare anche all'Italia il corretto approccio da adottare per garantire un equilibrio stabile tra concorrenza economica e sviluppo sostenibile. sostenibile. Il primo capo del disegno di legge sulla concorrenza oggi in discussione disciplina la materia energia e prevede l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Purtroppo però non dà seguito allo snellimento delle procedure per la realizzazione delle comunità di energia rinnovabile e di autoconsumo collettivo. Sappiamo benissimo quanto il costo dell'energia costituisca un fattore decisivo e strategico per la concorrenza economica di un sistema produttivo. Ci sembra per questo irragionevole non prevedere misure che massimizzino i benefici economici derivanti dalla generazione distribuita di energia elettrica e da un maggior supporto per l'autoproduzione energetica individuale e collettiva. Per questo noi di Alleanza Verdi e Sinistra rivediamo la necessità di accelerare la diffusione delle soluzioni contrattuali maggiormente utilizzate in Europa per i nuovi impianti a fonti rinnovabili con i contratti a lungo termine e contratti per differenza, di prevedere misure a favore dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche che per essere economicamente sostenibili devono autoconsumare almeno il 60-70 per cento dell'energia generata. Più che sfruttare questo disegno di legge come viatico per traghettare in modo deciso l'Italia verso la transizione energetica, la maggioranza in Commissione ha invece deciso di inserire e approvare un emendamento sgangherato e rischioso per aumentare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici, portandolo da 6 a 15 volt per metro. La materia è tecnica e complessa e francamente non può essere liquidata tramite un semplice emendamento, tanto più che questa mossa avventata della maggioranza sta mettendo in serio allarme i cittadini, le associazioni, gli esperti del settore e le comunità scientifiche. Per questo motivo abbiamo chiesto una seria e approfondita analisi, anche tramite un'indagine conoscitiva, ribadendo fra l'altro che nell'emendamento appaiono parametri tecnici che andrebbero illustrati in sede opportuna. La maggioranza in Commissione ha bypassato intenzionalmente questa richiesta, approvando questo rischioso emendamento. Su questo tema ci preme ricordare che innalzare il valore di attenzione per i luoghi di vita, dove si permane per più di quattro ore, risulta pericoloso per la salute umana e per l'ambiente. Anche al di sotto degli attuali *standard* di sicurezza, produce danni alla salute e riduce i livelli di benessere, soprattutto tra i soggetti vulnerabili, come bambini, donne in gravidanza, malati cronici, malati di tumore ed elettrosensibili. Alla maggioranza piace raccontare che in tutta Europa i valori dei campi elettromagnetici sono più alti. Si dimentica tuttavia che in Italia dal 2012 il fattore delle radiazioni dei campi elettromagnetici viene calcolato su una media di di 24 ore, anziché di sei minuti (come invece avviene in Europa), e che i sei minuti sono raccomandati dalla comunità scientifica. Il valore medio calcolato sulle ventiquattr'ore risulta così falsato, perché gli alti picchi registrati nella fascia diurna vengono facilmente compensati dai valori notturni bassissimi, perché ci sono pochi utenti attivi. Su questo punto la ricerca scientifica è molto chiara e il limite raccomandato, pari a 6 volt per metro misurato in sei minuti, è l'unico che garantisce il rispetto del principio di precauzione, evitando danni futuri. Non paghi di questo innalzamento dai 6 ai 15 volt per metro, il Governo ieri ha presentato un altro emendamento che aumenta il valore di intensità di campo magnetico e della densità di potenza, dando solo un'ora di tempo per subemendarlo. A quanto pare, questi temi sulla salute sono poco cari a questo Governo, che vanno a sommarsi a tutti quelli che stanno già pregiudicando la salute dei cittadini in Italia. Cito solo la pessima qualità dell'aria e le falde acquifere inquinate da sostanze perfluoroalchiliche L'ulteriore schiaffo che la maggioranza sta dando all'economia italiana scaturisce però dalla presunzione di voler modernizzare il nostro Paese puntando sul *made in Italy* e sulla forza lavoro dell'imprenditoria italiana, tutto l'opposto rispetto a ciò che invece fa con questo emendamento, con il quale si accontentano unicamente gli interessi dei colossi stranieri delle telecomunicazioni, perché questo è. Non esiste infatti in sé alcuna ragione per innalzare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici generati dalle radiofrequenze, se non quella economica di favorire i gestori delle telecomunicazioni, con sede all'estero, che intendono risparmiare sui costi delle infrastrutture dopo aver acquistato le licenze per il 5G. Il 62 per cento degli impianti in Italia non risulta attualmente espandibile al 5G. Con i valori attuali dei campi elettromagnetici servono quindi nuovi siti e quelli già esistenti vanno reingegnerizzati, il tutto per un costo stimato di 4 miliardi, a carico degli operatori radiomobili stranieri e a discapito delle aziende italiane, che potrebbero svolgere i lavori. Con questo emendamento, che vuole aumentare il livello a 15 volt per metro, si regalano quindi profitti miliardari alle multinazionali straniere. Con buona pace del *made in Italy*. Chiediamo di affrontare con serietà questo tema e auspichiamo che la maggioranza faccia oggi marcia indietro su questo argomento, accertando concretamente quali siano le ricadute dell'esposizione dei tessuti cellulari alle radiazioni e a radiofrequenze provenienti dall'intero campo elettromagnetico, prima di approvare il tutto. Abbiamo infine proposto, in materia di assegnazione delle concessioni sulle aree pubbliche, un ordine del giorno per assegnare almeno il 30 per cento di queste concessioni a piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero. La valorizzazione e la promozione di questi prodotti in linea con la normativa nazionale ed europea in materia favorisce sistemi di coltivazioni locali e sostenibili, garantisce la freschezza e la stagionalità dei prodotti e riduce l'inquinamento legato al trasporto della merce e alla necessità di *packaging*. Di tutto questo dispiace prendere atto. Chiudo il mio intervento ribadendo al Governo, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, la necessità di eliminare i vincoli normativi e burocratici che ostacolano ingiustificatamente la trasformazione ecologica di tutti i settori dell'economia

ci troviamo di fronte a un passaggio inconsueto che utilizza, più che legittimamente, uno strumento che è sempre stato visto come uno strumento della maggioranza per superare ostruzionismi, fino a ieri, probabilmente anche in questo momento e dopo, ci si lamenterà del fatto che non c'è abbastanza tempo e che i tempi sono ristretti. Chiedere a questo punto che non si possa fare gran parte della discussione generale non è particolarmente coerente con le accuse di volere stroncare la discussione, ma noi ci stiamo e tutto sommato potrebbe anche non dispiacerci di chiudere la discussione generale. generale. Non so cosa ne pensino i colleghi degli altri Gruppi di maggioranza, ma potremmo anche accettare di votare a favore della chiusura anticipata della discussione.

Grazie

del commercio sul suolo pubblico. Io penso - e ve lo dico in maniera molto chiara e sincera - che in questo caso abbiamo finalmente dato una mano a un settore che ha subito una crisi estremamente pesante, soprattutto nel periodo del Covid, perché da 180.000 esercizi si è passati, nel giro di un paio d'anni, a meno di 160.000. Si tratta

problematico e decisivo aver prorogato di un anno le attività che si svolgono all'esterno dei locali, soprattutto in un momento come quello attuale.

Questo nasce da ordinanze trasversali e finalmente si è trovato un punto fermo che va verso la tutela dei nostri centri storici, con la possibilità per i nostri sindaci di limitare alcune attività che non siano in linea con la programmazione turistica e con la loro valenza storica, artistica

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 18.0.106

queste sono occasioni in cui dobbiamo cercare di dare allo Stato tutti i poteri possibili per quanto riguarda alcune delle componenti imprescindibili per la salvaguardia della proprietà intellettuale

il livello dei campi elettromagnetici di cui ho parlato prima. In Commissione, tramite un emendamento del senatore Pogliese, approvato in quella sede, si è ritenuto di voler aumentare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici da radiofrequenza a quindici volt per metro, senza avviare un'accurata analisi preventiva e senza considerare il fatto che aumentare il valore di attenzione per i luoghi di vita, dove si permane per più di quattro ore, risulta un motivo di grande preoccupazione, visti gli accertati danni alla salute che può provocare. Da almeno vent'anni è dimostrato che l'esposizione alle radiofrequenze, anche al di sotto degli attuali *standard* di sicurezza, produce danni alla salute, all'ambiente e alla biodiversità e riduce i livelli di benessere nella popolazione, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, come i bambini, le donne in gravidanza, i malati cronici, di tumore e gli elettrosensibili. Parliamo di una materia molto tecnica e complessa che, per essere adeguatamente trattata, necessita di un congruo tempo di analisi e approfondimento, che abbiamo chiesto anche in Commissione. E non necessita di un frettoloso emendamento in un disegno che, invece di promuovere il *made in Italy*, come ampiamente sbandierato da questo Governo, si preoccupa di sfavorire sfacciatamente gli interessi dei colossi delle telecomunicazioni, tra i quali non figurano aziende italiane. E questo va a scapito delle aziende italiane. Chiediamo di affrontare con serietà la questione dei campi elettromagnetici e auspichiamo che questa Aula faccia oggi marcia indietro sull'argomento, consentendo invece di avviare un'indagine conoscitiva, strumento necessario per accertare quali siano le ricadute delle esposizioni dei tessuti cellulari aumentando il livello dei campi elettromagnetici. Alla maggioranza piace raccontare che in tutta Europa i valori dei campi elettromagnetici sono più alti. Ciò che non racconta è che in Italia, dal 2012, la misurazione delle radiazioni dei campi elettromagnetici viene calcolata su una media di ventiquattro ore anziché di sei minuti, come avviene in Europa, e che i sei minuti sono raccomandati dalla comunità scientifica. Non è difficile capire che, se il valore medio è calcolato

La ricerca scientifica è molto chiara e il limite raccomandato, pari a 6 volte per metro misurato in sei minuti, risulta il più consono per assicurare il rispetto del principio di precauzione e per tutelarci da danni futuri. Ci associamo quindi agli appelli della comunità scientifica, alle evidenze scientifiche e alle ricerche internazionali, chiedendo alla maggioranza di Governo un atto maturo e di buon senso, ritirando l'articolo. Aggiungo anche che, non paghi di questo innalzamento approvato in Commissione, ieri il Governo ha presentato un altro emendamento che aumenta il valore di intensità di campo magnetico e della densità di potenza, dando solo un'ora di tempo per subemendarlo. chiediamo quindi se in Commissione sia stata approvata una formula errata. Ce lo chiediamo e mi sembra che sia legittimo farlo. A maggior ragione chiediamo con forza di ritirare tutto l'articolo 10. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento che, peraltro, è identico al nostro precedente. E sollecito l'Assemblea e la maggioranza a valutare l'opportunità dell'applicazione del principio di precauzione, sempre consigliato nel momento in cui si parla di tutela della salute delle persone. Per aggravare la possibilità di mettere a rischio la salute delle persone con una decisione che pare tra l'altro anche poco ponderata, non essendoci stato un sufficiente confronto in Commissione,

di non mettere mano a questi limiti, per tutte le ragioni che ha ben spiegato prima la senatrice Floridia, per la tutela della salute dei cittadini del nostro Paese, 9a Commissione si sia fatta spregio dei pareri scientifici e vada ad innalzare vergognosamente dei limiti di legge che mettono a rischio la salute degli italiani. con quale coraggio il Presidente di quella Commissione abbia potuto mai permettere che si votasse e si portasse avanti una simile proposta. Per favore, lasciamo finire la senatrice. PIRRO *(M5S)*. Non tutti voi avete qualche nozione di scienza e di medicina. Non tutti voi sapete quanti e quali danni possono provocare i campi elettromagnetici, pur se nel nostro Paese di studi in tale ambito ne sono stati prodotti moltissimi. Mi domando se, come al solito, questa maggioranza abbia più a cuore gli interessi di pochi - e a volte non si capisce neanche di chi piuttosto che quelli dei cittadini del nostro Paese e soprattutto la salute dei cittadini del nostro Paese. Dovreste vergognarvi se non approvate questi emendamenti.

il motivo per il quale siamo contrari sia a questi emendamenti, sia all'articolo 10, consiste proprio nell'evitare situazioni di discussioni su tematiche scientifiche. Noi dobbiamo ai cittadini la serenità, soprattutto quando si utilizzano tecnologie come gli *smartphone* o tutto ciò che è legato alla transizione digitale. Abbiamo il dovere di dare certezza di far capire alle persone che ciò che noi decidiamo in termini di parametri, anche per la loro salute, viene fatto rispettando delle procedure e le indicazioni della Commissione europea. attribuendo tali decisioni non ad emendamenti che cascano sul Parlamento, ma ad autorità indipendenti che assumono le responsabilità in base alle loro prerogative, alla alla spiegazione di tipo scientifico e alla considerazione dell'equilibrio e dell'analisi fra concorrenza, innovazione tecnologica e tutela della salute. in corso, da tanto tempo, su questa tematica un dibattito in Italia, perché effettivamente, al di là della misurazione, c'è una differenza tra diversi Paesi europei. Allora, o ci si adegua e si difende il principio dell'adeguamento europeo oppure, se si introduce un qualunque numero tra 6 e 61, tra 06 e 61, si ha il dovere di spiegare qual è stata l'analisi, qual è la valutazione di impatto e sulla base di quale spiegazione scientifica, tecnica, economica e concorrenziale

si alimentano speculazioni, incertezze e la preoccupazione e la paura che le decisioni che prendiamo sotto il profilo pubblico non siano dettate da un rigoroso e attento esame di tutte le implicazioni, ma siano l'emendamento cascato sul Parlamento ad opera di chi è stato più capace, fra i diversi operatori, di convincere qualcuno. Questo è sbagliato perché alimenta le incertezze. Noi abbiamo presentato qualche settimana fa un disegno di legge nel quale proponiamo l'istituzione, come in Francia, di un'Agenzia per le frequenze, che unisca le competenze, in parte di Agcom, del Ministero dello sviluppo economico e del *made in Italy* e delle ARPA. A proposito di concorrenza, voi avete dimenticato una segnalazione dell'Autorità *antitrust* di qualche anno fa che sosteneva che le possibili e diverse misurazioni delle ARPA regionali potevano avere un impatto concorrenziale nei diversi pezzi del territorio italiano. Quindi, non solo non avete introdotto una norma, assicurando un percorso trasparente e convincente per tutti, ma non avete neanche risolto il tema concorrenziale che avrebbe dovuto legare questo emendamento del disegno di legge concorrenza. Per queste ragioni esprimo voto contrario perché si sceglie un metodo che alimenta le incertezze, le paure e semplicemente propone come strumento di decisione politica

Signor Presidente, volevo dire, tramite lei, alla senatrice Pirro che non mi vergogno di votare contro gli emendamenti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato sul tema dei campi elettromagnetici. Non mi vergogno perché, avendo fatto la Presidente della Commissione trasporti, ho potuto approfondire il tema del 5G in modo molto serio. Lo dico anche al collega Licita, che stimo, ma questa volta ha detto cose lontane anni luce da ciò che penso io ed è stato approfondito e sviscerato da tutte le latitudini, compreso l'Istituto superiore di sanità. Allora, bisogna capirci: un tema è rendere il nostro Paese competitivo e da questo punto di vista noi abbiamo, nel tema dell'innovazione digitale e tecnologica, un dovere in più di fare la nostra parte; un altro tema è istituire nuovi strumenti di garanzia, come Autorità, ma fatemi dire che in questo Paese ce ne sono anche troppi. per verifiche e analisi che funzionano in tutto il globo e che sono state sviscerate a pieno titolo all'interno delle Commissioni competenti, credo non ci sia bisogno di istituire nuove agenzie e nuove Autorità. pensiero. Quello che soprattutto ci tengo a dire è che non accetto lezioni di moralità e di etica da parte di una forza politica, il MoVimento 5 Stelle, che Lasciamo intervenire la collega, per favore. PAITA

contro l'innovazione tecnologica in uno strumento come questo. Per cui non solo non mi vergogno, ma chiedo anche che ci sia un po' di serietà in quest'Aula quando si parla di questioni veramente importanti per le nostre imprese e per i nostri cittadini. *(Applausi)*.

una volta l'energia elettrica si trasportava coi tralicci, e adesso abbiamo scoperto che è meglio farla passare sotto terra piuttosto che in alto, perché determina delle ripercussioni su quelli che abita nelle vicinanze.

europei. A coloro che mi hanno scritto e mi hanno contattato - anche loro contrari a questa misura, anche persone che affermavano di avere conoscenze di siffatto tipo - ho chiesto se esiste un solo studio

dalla senatrice Aurora Floridia, quando ha detto che in questo provvedimento si fa riferimento alla media giornaliera anziché a quella puntuale, spiegando che di notte c'è un traffico inferiore, tipicamente quello dei nostri telefonini, e dunque la media si abbassa. È vero, ma la notte, largheggiando, dura quanto il giorno. In realtà la notte civile dura un terzo o un quarto della giornata. Ma, se supponiamo che sia la metà, vorrebbe dire che tuttalpiù siamo ancora più di due volte sotto il limite europeo

I telefonini, lo strumento che maggiormente contribuisce al fenomeno dei campi elettromagnetici, funzionano un po' come noi con la nostra voce: più il segnale è basso, più il telefonino trasmette un segnale potente. Questa è la ragione per cui, quando andiamo in montagna, dove c'è un segnale basso o è assente, il nostro telefonino cerca di trovare una connessione, consuma molto di più la batteria, che quindi si esaurisce più rapidamente. Pazienza. Il punto è che, se il campo elettromagnetico è più basso, il nostro telefonino trasmette un'intensità più alta e, siccome l'intensità del campo elettromagnetico è inversamente proporzionale alla distanza, il nostro telefonino, che teniamo a un centimetro dal cervello, è enormemente più pericoloso di un'antenna che come minimo sarà a una cinquantina di metri di distanza, cioè sarà 5.000 volte più distante dal nostro cervello di quanto lo sia il telefonino. Pertanto, con i limiti così bassi i nostri telefonini trasmettono intensità maggiore a un centimetro dal nostro cervello; mentre, con un innalzamento dei limiti, sarà possibile avere un maggiore equilibrio. Dice molto bene l'articolo 10 nel suo testo, che comunque bisogna portare avanti degli studi, osservare e vedere quali sono gli effetti. Il confronto fra le opinioni è fondamentale in tutti i campi scientifici, non solo sui campi elettromagnetici. È su questa base che il Governo ha proposto questa norma e su questa base è stato presentato un emendamento ed è per questo che voteremo contro gli emendamenti soppressivi.

solo per far presente, fra le varie considerazioni, che vi è uno Stato nostro confinante che viceversa applica il principio di precauzione mettendo in secondo piano l'aspetto economico concorrenziale rispetto all'aspetto della tutela della salute e questo Stato è la Svizzera. La Svizzera, anziché peggiorare questi limiti, li ha innalzati, mentre non li stiamo abbassando, mettendo a rischio la salute dei cittadini. C'è quindi qualcuno che ragiona e legifera partendo da presupposti diversi.

questa leggenda della salute che viene violata solo perché si innalzano dei valori elettromagnetici, quando siamo circondati

al pericolo per la salute umana, con studi scientifici che lo dimostrano, mi ricorda tanto gli studi scientifici fatti per decenni per evitare un'opera, l'alta velocità

dei cittadini ignari di quanto noi stiamo facendo. Forse le forze politiche, invece di sollecitare quelle paure, dovrebbero dare risposte

chiediamo di assegnare almeno il 30 per cento di queste concessioni a piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli alimentari provenienti da filiera corta a chilometri zero. La valorizzazione e la promozione di questi prodotti, in linea con la normativa nazionale ed europea in materia, favorisce sistemi di coltivazioni locali e sostenibili, garantisce la freschezza e la stagionalità dei prodotti e riduce l'inquinamento legato al trasporto della merce e alla necessità di *packaging*. Ciò che intendiamo promuovere è una nuova economia, che possa essere circolare, equa, ambientalmente sostenibile e maggiormente attenta a favorire nuovi stili di vita. Quindi, chiedo che questo ordine del giorno

6.20, si parla del *vertical farming*. Vorrei sottolineare che il MoVimento 5 Stelle già nella passata legislatura era pienamente consapevole dell'utilità di eliminare da questo ambito le fasi di asciugatura e lavatura. Quindi, non so perché il mio emendamento non sia stato

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

della confusione che spesso si fa fra il concetto di concorrenza, il concetto di mercato e l'antitrust. Sono consapevole che questa è una misura che è stata suggerita dall'Autorità antitrust,

nel settore delle comunicazioni elettroniche di discriminare, di fare offerte selettive di prezzo, tra le altre cose, in base alla provenienza dell'operatore di riferimento. Non si possono cioè più fare delle offerte selettive in funzione dell'operatore con il quale attualmente il consumatore è impegnato. Da un certo punto di vista questa effettivamente è una misura che impedisce ad alcuni operatori di fare offerte favorevoli soltanto ai clienti dei concorrenti che si vogliono acquisire. tratta di una pratica di sconto selettivo che, dal punto di vista della teoria economica, è sempre stata giustificata, sotto il profilo antitrust, quando questo comportamento di sconto è associato ad una posizione di dominanza individuale o collettiva del soggetto che fa lo sconto. Cioè il soggetto che fa lo sconto selettivo soltanto ad alcuni clienti del concorrente ha un vantaggio in più rispetto al concorrente, che è quello di potersi permettere di finanziare in perdita determinate offerte, mentre il concorrente non può fare la stessa cosa, d'altra parte, con i clienti del concorrente che gli vuole rubare i propri clienti; non c'è una reciprocità di reazione. Quando questa reciprocità di reazione non c'è, vuol dire che c'è una dominanza e che quindi è la dominanza, di fatto, a esercitare un potere di mercato e a rendere anti-concorrenziale lo sconto selettivo. Nella teoria economica antitrust, questa clausola della nazione più favorita o *matching clause*. Invece, quando non c'è una dominanza, l'idea che io non possa fare un'offerta ai clienti del mio concorrente si scontra con l'idea che anche il mio concorrente potrebbe fare la stessa cosa nei confronti dei miei clienti. Allora sarà il mercato, nella razionalità degli operatori, a stabilire quali sono gli sconti di equilibrio sul mercato. Noi invece qui stiamo introducendo un principio per cui, non potendo più fare sconti selettivi, o si farà lo stesso sconto per tutti i clienti o non lo si farà. Ma, se non lo si farà, alla fine i prezzi si alzeranno. Quindi questa norma, scritta così, può finire per introdurre incentivi ad incrementare il prezzo medio per i consumatori finali e non a favorirlo, a meno che non aveste scritto nella norma "nel caso in cui esiste una posizione dominante individuale o collettiva". Ma d'altra parte, se ci fosse una posizione dominante o collettiva,

una over-regolazione su questioni che dovrebbero essere lasciate alle dinamiche di mercato o alle norme esistenti, perché già tutta la normativa del codice delle comunicazioni attribuisce all'Agcom la possibilità di vietare forme di discriminazione

Io sono pronto a scommettere con voi che, se questa norma funziona, fra un anno tutti i consumatori di tutti gli operatori avranno prezzi medi più alti. in un mercato che ha dei prezzi molto bassi, potrebbe essere uno strumento di sostenibilità del mercato. Ma allora non chiamiamolo uno strumento di concorrenza e di discriminazione; è uno strumento che serve ad evitare una concorrenza distruttiva e predatoria,

su un argomento già dibattuto più e più volte in quest'Aula: parliamo dell'esercizio della professione di odontoiatria in forma societaria. In Italia è ancora possibile per un gruppo di imprenditori aprire una clinica, perciò dare priorità a quella che è un'attività meramente commerciale a discapito della qualità e del rispetto della salute dei pazienti. Con il nostro emendamento noi chiediamo al Governo la massima attenzione, anche perché siamo sicuri che il Governo e la maggioranza abbiano a cuore la salute dei pazienti e mettano sicuramente in prima linea la qualità del servizio e non il profitto, che spesso è invece il faro che guida

per porre rimedio a questo, c'è una via ben chiara: dare la possibilità ai professionisti che operano in questo settore, cioè gli odontoiatri, che si vogliono unire in forma societaria, secondo la formula della società tra professionisti, perciò senza l'intervento prevalente del capitale. In

primo obiettivo di tutti i presenti in quest'Aula, anche se a volte ci viene il dubbio che non sia propriamente così. In questo caso ci troviamo di fronte a a discriminazioni che vengono effettuate a volte dalle compagnie assicurative, nello specifico per quanto riguarda le assicurazioni sanitarie integrative, in quanto la maggior parte dei nuovi contratti prevede che le coperture assicurative e il rimborso delle prestazioni vengano erogati ai soggetti esclusivamente se si rivolgono a centri direttamente convenzionati con la compagnia assicurativa. Questo di sicuro comporta uno sconto e una riduzione dei costi a carico dell'assicurazione, ma non sempre si traduce in un'adeguata copertura dei diritti del paziente/cliente dell'assicurazione. Questo avviene perché non sempre ci sono centri convenzionati nelle immediate vicinanze o facilmente raggiungibili dai cittadini che hanno stipulato queste polizze; in secondo luogo, per le che spiegava il collega Lorefice poc'anzi, si tratta a volte di grandi centri dove non è garantita una prestazione ottimale e l'uso di materiali ottimali:

un paziente non possa rivolgersi ad un medico di propria fiducia, ma sia obbligato a rivolgersi esclusivamente al centro convenzionato. Sulle polizze assicurative sanitarie integrative si potrebbe dire tantissimo; non voglio aprire quel capitolo in questa sede, ma quantomeno la tutela della salute (e quindi del rapporto fiduciario) dovrebbe essere un faro per noi, anche perché la nostra polizza assicurativa integrativa, per esempio,

che lo stesso diritto fosse garantito per legge a tutti i cittadini italiani, ponendo eventualmente un tetto che prefiguri il rimborso a carico del cittadino in misura pari a quello che sarebbe stato il costo per la compagnia assicurativa della medesima prestazione effettuata in un centro convenzionato. Non si chiede che paghino di più; si chiede che paghino la stessa cifra, ma che non violino il rapporto di fiducia tra cittadino e medico.

Signor Presidente, per il suo tramite mi rivolgo anche al Governo e mi permetto sommessamente di ricordare che questo tema è stato trattato

è stato accolto con la formula piena, impegna il Governo nel primo provvedimento utile a intervenire sulla disciplina della forma societaria delle cliniche odontoiatriche, prevedendo che queste possano esercitare nella forma di società

il Governo in questo modo smentisce se stesso e anche la maggioranza. Vi rendete conto di quello che fate? Avete accolto un ordine del giorno con il preciso impegno che al primo provvedimento utile avreste provveduto a dare seguito all'impegno preso e ora smentite voi stessi. Fate capire a noi e agli italiani dove volete andare, qual è la vostra onestà intellettuale, la vostra serietà.

non rispettano un impegno preso in questa sede, che è il Senato della Repubblica.

Se vi ricordate, in quell'occasione all'articolo 1, commi 5 e 6, sono stati modificati i poteri dell'Autorità *antitrust*, dell'Autorità *antitrust*, che oggi può imporre rimedi o accettare impegni strutturali e comportamentali di imprese all'interno di una procedura che è o di intesa o di abuso di posizione dominante o come rimedi in operazioni di concentrazione. In questa norma, invece, è stato introdotto un principio che non c'era nell'ordinamento, ossia la possibilità che l'Autorità *antitrust*, dopo aver lanciato un'indagine conoscitiva, laddove riscontri problemi anticoncorrenziali che non sono né di abuso di posizione dominante, né di cartello, imponga comunque rimedi alle aziende.

e cioè che in questi mercati vi sia una posizione dominante individuale o collettiva, perché, se non c'è una posizione individuale o collettiva dominante, significa che stiamo dando il potere all'Autorità *antitrust* di intervenire indipendentemente da distorsioni *ex ante* del mercato, situazione che potrebbe comportare elementi essi stessi distorsivi. facendo riferimento alla legislazione a cui quella norma si ispira, cioè la legislazione *antitrust* del Regno Unito, proponiamo che si espliciti

nel diritto *antitrust* italiano, perché significa che facciamo fare all'Autorità *antitrust* politica industriale: l'Autorità apre un'indagine conoscitiva, vede che qualcosa non funziona e impone rimedi, ma questo dovrebbe farlo chi è responsabile di politica industriale. Altra cosa è se invece, coerentemente con la legge n. 287 del l'*Antitrust* agisce nel contesto di una posizione dominante individuale o collettiva, perché lì esercita i propri poteri e si collega al concetto di potere di mercato. Per questo chiedo una riflessione su questo emendamento, anche perché quella è una norma che modifica paradossalmente i poteri dell'Autorità *antitrust* solo in un settore, cioè in quello dei trasporti. Evidentemente, in futuro questo avverrà anche in altri settori e, dal punto di vista della coerenza del diritto *antitrust*, effettivamente è un'anomalia che è stata introdotta. quindi una riflessione da parte dei relatori per cercare di ricondurre nell'alveo dei tipici poteri di un'Autorità *antitrust* conforme al diritto europeo anche queste nuove prerogative che sono state introdotte con il decreto

si conferisce all'Autorità *antitrust* l'incarico di autorità designata per l'attuazione della regolamentazione europea denominata Digital markets act. Come sapete, della nuova disposizione di regolamentazione europea che va a disciplinare in modo nuovo, quindi anche innovativo rispetto alla legge *antitrust*, *antitrust*, le questioni relative ai cosiddetti *gatekeeper*, cioè le grandi piattaforme *online* attive in tutta una serie di settori e che sono oggi oggetto di una nuova regolamentazione pro concorrenziale. Quello che accadrà, e che evidentemente accade, è che questa è una regolamentazione particolare, perché riguarda le piattaforme. Come sapete, le piattaforme *online* sono di varia natura. La Commissione europea ha individuato un certo numero di di *gatekeeper* che sono oggetto di particolare regolamentazione e ovviamente sono attivi in tanti settori e in tanti mercati diversi. Tipicamente, guardando alla legge *antitrust* italiana, ma anche alle normative che hanno introdotto la legislazione di settore, c'è sempre un principio che viene previsto dalla normativa italiana e cioè che quando un'Autorità *antitrust* prende una decisione che riguarda un settore, deve acquisire il parere di un'*Authority* indipendente di settore di regolamentazione, proprio per cercare di avere più informazioni. Con l'emendamento semplicemente reintroduciamo questo principio anche a proposito del Digital markets act, per cui quando ci dovesse essere un intervento che riguarda situazioni ad per piattaforme *social*, allora si direbbe all'Antitrust di acquisire anche il parere dell'Agcom; quando c'è un tema che riguarda l'autorità dell'energia e i contatori, gli si dice acquisire, prima di prendere una decisione, anche il parere dell'ARERA; quando c'è un tema che riguarda l'autorità dei trasporti, gli si dice di acquisire il parere dell'autorità dei trasporti o, nel caso di dati o algoritmi, anche quello in particolare del Garante. Stiamo semplicemente cercando di restituire di restituire a un principio di designazione italiana, e quindi di applicazione del diritto europeo, una piccola *golden rule* che semplicemente attribuisce alle diverse *Authority* una capacità di coordinamento e di confronto, acquisendo pareri, semplicemente per permettere di valutare non soltanto i profili strettamente concorrenziali, ma anche quelli più strettamente legati alle esigenze della regolamentazione. Si tratta di una piccola cosa e sinceramente mi auguro che almeno in questo i relatori e il Governo possano seguirci.

intervengo per ricordare che oggi a Padova comincia questo incredibile processo nel quale lo Stato stabilisce di decidere se una famiglia è una famiglia. un processo che prevede che i giudici entrino nelle case di mamme e bambini che sono cresciuti insieme e di persone che hanno stabilito un legame d'affetto. Sulla base di una qualche legge, si vorrebbero togliere dei cognomi a dei bambini e separare quello che l'affetto ha creato e quei nuclei familiari, tutto in un Paese nel quale ci si riempie la bocca dell'assenza di nuovi nati e dell'importanza della famiglia. Io credo che sia un sopruso un sopruso insopportabile. Penso che tutta l'opinione pubblica e - temo - anche le opinioni pubbliche di altri Paesi guarderanno a questo processo di Padova come a un grande arretramento dal punto di vista dello Stato di diritto per un Paese che si vanta di essere la culla del diritto. Io penso che sia veramente un momento

Abbiamo oggi portato avanti due bellissime iniziative: una, questa mattina, al Ministero della salute con il ministro Schillaci e l'Intergruppo parlamentare di cui mi onoro di essere presidente, insieme al collega della della Camera Roberto Pella e a tante colleghe e colleghi che sono qui in Aula di tutti i Gruppi politici, che ringrazio moltissimo; nel pomeriggio, si è svolto un importante convegno, a cui ha partecipato anche il presidente Zaffini della 10a Commissione, che ringrazio moltissimo,

fatto una legge sul diabete e sulla celiachia. Mi auguro che tante altre iniziative possano lavorare soprattutto sulla cultura della prevenzione, che è quello che serve nel nostro Paese. **Atti e documenti,